L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

chiusa la votazione. **Il Senato non approva**.

Per favore, calma. Adesso i Segretari riferiranno alla Presidenza; ciascuno faccia il suo mestiere.

Dichiaro chiusa la votazione. **Il Senato non approva**.

l'ordine del giorno G2.100, che sta a dimostrare come noi, a differenza di quanto in quest'Aula è stato insinuato,

tanto declamato come elemento di garanzia per la riuscita dell'operazione, ha invitato il Parlamento a consentire l'autorizzazione delle due discariche che hanno già ottenuto la valutazione d'impatto ambientale positiva all'interno dello stabilimento.

gli emendamenti all'articolo 2,

su moltissimi ordini del giorno alla stessa risposta sia da parte del relatore, che del rappresentante del Governo: no o invito al ritiro. Vorrei capire se il no del relatore e del Governo è un no che entra nel merito dei singoli emendamenti

fino alle parole «da euro», con parere positivo di relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione.

il decreto-legge che stiamo esaminando. È davvero inaccettabile trincerarsi dietro ad un no, che non ha nessun tipo di motivazione. L'errore di prima ha fatto vedere la modalità di voto di questa maggioranza, che non entra nel merito della qualità degli emendamenti, ma vota secondo una regia, che gli italiani devono capire, e secondo interessi che non sono quelli dei cittadini.

a valutare l'opportunità di considerare strategico il processo di riqualificazione», espungendo le parole «a puntare sul».

Il decreto prevede lo stanziamento di 90.000 euro all'anno nel triennio per gli assegni agli ispettori dell'ISPRA,

Dichiaro chiusa la votazione. **Il Senato non approva**.

ahimé, la deroga al Patto di stabilità alla Regione Puglia per ben 40 milioni di euro.

la riduzione della spesa rilevante del Patto di stabilità per 300 milioni di euro a beneficio di tutte le Province. Sull'emendamento c'è stato il parere negativo della 5a Commissione e ne abbiamo chiesto la trasformazione in ordine del giorno. Vedete, le Province italiane stanno tutte soffrendo.

prima la soppressione e poi il riordino delle Province. Qualche giorno fa anche il TAR del Lazio si è pronunciato, di fronte a un ricorso della Provincia di Genova, e ha bocciato sostanzialmente i criteri e l'entità dei tagli alle Province. Il Governo da poco ha fatto un disegno di legge costituzionale che vuole svuotare le Province, ma queste esistono, come esistono le strade provinciali, gli istituti superiori

hanno beneficiato poco o per nulla. Infatti, gli enti che hanno beneficiato e beneficeranno di questo decreto sono soprattutto gli enti spendaccioni che lo scorso anno hanno avviato gli appalti senza avere le necessarie coperture finanziarie, mentre gli enti virtuosi che hanno voluto rispettare il Patto di stabilità hanno delle risorse da poter spendere in appalti dando lavoro alle imprese e, quindi, creando occupazione. è un ordine del giorno che darebbe lavoro e, quindi, occupazione a molte imprese e lavoratori.

ad interpretazioni non corrette, che stiamo parlando di una deroga all'utilizzazione di risorse statali già assegnate alla Regione Puglia; si tratta ovviamente di una deroga al patto di stabilità

Il tema ci è noto ed è ovviamente condivisibile; ma parliamo di un tema

dello svuotamento di risorse in capo alle Province, in presenza di una continuità di funzioni che tutte le Province del nostro Paese stanno continuando ad esercitare, nelle more dell'applicazione di una riforma costituzionale. Il tema però ci sembra estraneo all'oggetto del decreto, e comunque ci rimettiamo al Governo.

Signora Presidente, nell'ultima fila in alto, nel Gruppo dei grillini, c'è un posto vuoto e un segnale verde.

senatore Scilipoti ha segnalato, i senatori Segretari hanno preso nota ed hanno verificato. Per favore, i senatori Segretari hanno già verificato e preso nota...

non può essere, però, a senso unico il fatto che se un altro collega indica un'altra cosa si senta dare del buffone.

impegnare il Governo «ad adottare le opportune iniziative (...) allo scopo di permettere alle province, che pur disponendo delle necessarie risorse non hanno avviato lavori nel corso del 2013 per rispettare i limiti imposti dal Patto di stabilità interno, di riprendere le opere programmate», in quanto chi ha rispettato il Patto, e per rispettarlo non ha dato il via alle opere, viene impedito nel farlo anche successivamente. Non si chiedono degli stanziamenti: si chiede una rimodulazione, in modo che le Province virtuose possano riprendere quelle opere che sono state sospese per garantire quella virtuosità. A questo aggiungiamo che, oltre ad una sentenza della Corte che ha dato torto al Governo perché è

il problema è che non c'è; forse qualcuno può dirmi che non c'è uno stretto nesso rispetto alla materia, ma nel decreto si parla di Patto di stabilità.

in condizioni normali avrei atteso la fine della seduta, anche per non esacerbare gli animi, ma poiché il senatore Calderoli ha avuto modo di muoverci un rilievo sulla reciprocità della correttezza

l'accortezza di scusarsene. A questo punto noi non ci stiamo a essere continuamente etichettati come

sia assicurata per un verso dal processo verbale delle sedute, di cui all'articolo 32 del Regolamento, e per altro verso dalle riprese del servizio televisivo del Senato

Mi chiedo però, signora Presidente, se questo possa avvenire quotidianamente

ai senatori quale televisione, e perché, è stata autorizzata

costantemente osservati, alle nostre spalle, da telecamere e macchine fotografiche che ovviamente riproducono a loro piacimento la nostra corrispondenza.

vorrei rispondere al senatore Palma: la televisione che è qui da diversi giorni è un *service* danese di cui non ho adesso il nome ma potrò fornirlo grazie agli Uffici - che ha chiesto l'autorizzazione a fare le sue riprese. Preciso altresì che il video di un momento particolarmente acceso della seduta di ieri non è stato prodotto da questo

gli emendamenti e gli ordini del giorno che facevano riferimento al commissario straordinario, che si possa trovare un modo per ripristinare la figura del Garante come figura di terzietà.

Va in questa direzione anche l'impegno cui abbiamo chiamato Governo, commissario e subcommissario nel relazionarsi in tal modo con la comunità locale e anche nel relazionarsi semestralmente con il Parlamento, rendicontando l'attività svolta sia nelle funzioni commissariali sia - specificamente - nelle funzioni precedentemente assegnate al Garante.

positivo di relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione.

Grazie,

seppure in presenza di una situazione difficile, il sottoscritto ha ritenuto di dover dare fiducia al loro operato e ai loro progetti. il settore della siderurgia è strategico per il nostro Paese, quindi è giusto compiere ogni sforzo perché possa essere rilanciato, purché in sicurezza. Ci auguriamo inoltre che l'approvazione di questo provvedimento serva per monitorare l'attività del commissario e del subcommissario ma, soprattutto, l'attività dell'industria perché - lo ripeto - è importante per la città di Taranto ma altrettanto importante e, forse, ancor di

Signora Presidente, colleghi senatori, uno scrittore meridionale, parlando dalla sua terra, si esprimeva con queste parole: «Per chi ci è nato, dura poco l'allegria di sentirsi seduto sull'ombelico del mondo. Subentra presto la sofferenza di non sapere districare, fra mille curve e intrecci di sangue, il filo del proprio destino». È una riflessione che, a mio parere, ben si coniuga con la storia di Taranto e, dunque, dell'Ilva. Perché Taranto, nell'immaginario di molti, è l'Ilva. Da molti mesi a questa parte la cronaca non ha dato tregua a questa bellissima città, costretta a subire l'incalzare delle inchieste e delle ordinanze della magistratura: dagli arresti dei Riva e dei loro dirigenti, passando per il sequestro degli impianti dell'area a caldo e, successivamente, del prodotto finito e semilavorato; dall'ordine di custodia cautelare per il presidente della Provincia di Taranto, fino al maxisequestro del capitale della famiglia bresciana La questione dell'Ilva è diventata così oserei dire finalmente, una questione nazionale. E non solo perché quello di Taranto è il più grande impianto siderurgico italiano uno dei più grandi d'Europa, ma soprattutto perché lì, in quel territorio, in quella parte di Puglia, quella fabbrica rappresenta l'anima dell'industria italiana, ma al contempo rappresenta rappresenta e ha rappresentato una rottura radicale della coesione sociale, della sostenibilità ambientale e del diritto alla salute e alla vita di un'intera comunità. Vedete, cari colleghi, l'Ilva di Taranto vanta molti *record*, alcuni positivi, tanti negativi. È il cuore della siderurgia italiana (è vero), capace di produrre fino a 10,5 milioni di tonnellate di acciaio che danno da vivere a circa 40.000 addetti tra diretti e indiretti, ma che possono anche far morire, perché purtroppo (anche questo è vero) è stata per troppi anni il maggior produttore nazionale di diossina, di polveri sottili e di altre sostanze tossiche, che hanno fatto della perla dello Ionio la città più inquinata d'Italia e presumibilmente d'Europa. la magistratura ha spesso parlato di disastro ambientale, dando nome e cognome ai responsabili: innanzitutto la famiglia Riva e, con loro, i massimi dirigenti che si sono succeduti in questi anni alla guida di questa società; responsabili di aver creato un danno ambientale incommensurabile, di aver generato quel cosiddetto sistema Ilva talmente pervasivo da lasciar immaginare una sorta di sudditanza psicologica di un intero territorio verso quella famiglia; sudditanza spesso alimentata da un non più sopportabile vero e proprio ricatto occupazionale e degenerata, in alcuni casi, in colpevoli comportamenti omissivi e conniventi all'interno di quel sistema che la stessa magistratura ha avuto il merito di svelare nelle sue pieghe più anguste attraverso le inchieste giudiziarie. Faccio questa premessa per dire che la Puglia per anni ha subito crimini ambientali e forme di colonialismo economico in un quadro di sciatteria che hanno cercato di trasformarla in una sorta di «territorio a perdere», in una terra in cui la grande industria ha avuto la licenza di violentare le identità ambientali e produttive (penso all'agricoltura ma anche alla pesca, con in cima la arcinota mitilicoltura di Taranto). Il decreto-legge in esame, il terzo in meno di un anno, nato inizialmente per commissariare l'azienda dopo il disimpegno evidente del gruppo Riva, si è via via trasformato in una sorta di abito cucito su misura, da questo Governo e da questa maggioranza, per limitare al minimo gli interventi di riambientalizzazione di quegli impianti previsti dall'AIA. In questa direzione, quest'Aula oggi si accinge ahimé a firmare questa ennesima cambiale in bianco, che ancora una volta metterà una pesante ipoteca sul destino di quella fabbrica, dei suoi lavoratori, ma anche di quel territorio e di quel sacrosanto diritto alla salute dei cittadini tarantini e pugliesi. Noi come parlamentari del Gruppo Misto-SEL, e anche io come parlamentare eletto in quella terra di Puglia, avevamo chiesto a questo Governo maggiore coraggio nell'affrontare una vicenda - è vero - complessa; avevamo chiesto di adottare scelte che fossero finalmente innovative sotto il profilo economico e anche sociale e ambientale (esattamente quello che si aspetta tutta la comunità ionica), comprese coerenza e continuità con il lavoro svolto dal 2005 in poi dal Governo regionale pugliese e da quella Assemblea legislativa, tantissimi provvedimenti legislativi innovativi rispetto ai quali il Governo nazionale si è puntualmente dimostrato avverso. In Parlamento, invece, si è scelta un'altra strada: quella di depotenziare, e dunque peggiorare, un decreto-legge entrato in Commissione alla Camera in un modo, e con un obiettivo ambizioso, ed uscito in un altro, finendo nuovamente per dare seguito solo a quei «bassi istinti» del capitalismo nostrano. Qui in Senato si è fatto ancora peggio: nonostante le tante sollecitazioni ricevute nelle tante audizioni svolte in Commissione (anche in trasferta in terra pugliese) si è avanzata la richiesta - grave, a nostro parere, ma non nuova nella prassi di questa maggioranza di chiedere il ritiro di tutti gli emendamenti al decreto, palesando così la totale indisponibilità a qualsiasi modifica o contributo migliorativo ed a difesa esclusiva della proprietà. Ci sono stati accolti solo pochi ordini del giorno, peraltro con una riformulazione proposta dal Governo e con un dispositivo che consentitemi di definire ridicolo. Penso ad esempio a quello che abbiamo fatto in ordine alla cancellazione definitiva della figura del Garante, istituita dalla legge n. 231 del 2012 del Governo Monti, quale figura terza e di garanzia incaricata di controllare che all'Ilva, gestita all'epoca direttamente dai Riva, si applicasse rigorosamente l'AIA rilasciata dal Ministero dell'ambiente. Lo abbiamo fatto finendo per confermare il trasferimento dei compiti del Garante - e questa è la vera innovazione - al commissario Enrico Bondi, già amministratore delegato della stessa azienda e, quindi, rappresentante nominato da quella stessa proprietà di cui dovrebbe controllare affidabilità e correttezza. Insomma, per dirla tutta: si è fatto finta di cacciare i Riva dalla porta perché inaffidabili per poi farli rientrare dalla finestra e metterli comodi! Noi abbiamo sostenuto altro e abbiamo chiesto, ad esempio, che non si peggiorasse il decreto come si è tentato di fare e e come ci aveva chiesto anche ampiamente l'ISPRA, visti i ritardi accumulati dall'azienda, che non si sforasse il limite del dicembre del 2015, imposto dal provvedimento licenziato dall'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini, nello scorso Ma abbiamo visto di più: abbiamo visto tentativi emendativi con i quali abbiamo tentato di concedere ai Riva di costruire e gestire discariche in barba ad ogni procedura di valutazione d'impatto ambientale. A questo punto, cari colleghi,

chi vigilerà sui tempi e sulle modalità? Ovviamente lo dovrà fare il dottor Bondi! E in quale veste? In quella di commissario che controlla l'affidabilità della proprietà e del suo *management* oppure in quella di curatore degli interessi della famiglia Riva? Presidente,colleghi, noi siamo fortemente preoccupati della eventualità che la proprietà di Ilva continui nell'atteggiamento di sempre: vale a dire quello di privatizzare e mettere in cassaforte gli incassi e socializzare invece le perdite e gli investimenti necessari alle opere di ambientalizzazione dei processi produttivi, portandoli a carico della collettività e della finanza pubblica procrastinarne *sine die* la effettiva e completa realizzazione. Ma siamo altrettanto preoccupati che continui ad esserci una parte della politica che si rifiuta di vedere quanto è accaduto nell'ultimo trentennio a Taranto e che continua a dimostrarsi, mi si passi il termine, flessibile. Sappiamo bene anche noi che il nostro Paese non può fare a meno della siderurgia e non può dimostrarsi superficiale

Che i figli di quella terra non continuino a vivere con una spada di Damocle sulla propria testa e sulla propria salute. Che le aziende dell'agroalimentare o del turismo jonico, solo per fare due esempi, non continuino ad essere violentate nella loro volontà di investire

Astensione come segnale politico chiaro, che giudica questa un'altra occasione persa, perché ad un buon proposito si è fatto seguire un atteggiamento lobbistico di modifica del testo, a sola protezione della stessa proprietà di sempre

garantire il lavoro a migliaia di operai, la conservazione di una grande realtà industriale e, al contempo, la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori è compito di un Governo che si rispetti ed è quello che dovrebbe fare questo decreto-legge. Esso prevede la nomina di un commissario e di un subcommissario con la prerogativa di rendicontare al Ministro dell'ambiente, al Ministro dello sviluppo economico e alle Commissioni parlamentari. È previsto il potenziamento degli organi di controllo ISPRA e ARPA nonché l'implementazione dei controlli sanitari ed epidemiologici. Certamente tutto questo è un grande sforzo e un grande impegno. Non siamo certi Non siamo certi che tutto questo si realizzerà nel migliore dei modi, né siamo certi che non si potesse fare di più. Ma abbiamo certamente il dovere di provvedere.

Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, nonostante le analisi approfondite e le tante audizioni sull'Ilva di Taranto, nonostante la costosa missione organizzata per costatare le criticità ambientali del sito, su proposta del Governo e con l'accordo della maggioranza, al Senato è stato precluso intervenire sul decreto-legge per correggere alcune evidenti lacune. È l'ennesima occasione mancata. Il Governo, per l'ennesima volta, si è appellato all'urgenza snaturando il ruolo del Parlamento e costringendoci, ancora una volta, a licenziare un provvedimento che, lo sappiamo tutti, non sarà risolutivo. apprestiamo, dunque, a varare l'ennesimo pasticcio all'italiana. Che senso ha parlare di urgenza quando da oltre quarant'anni perdura l'inquinamento di Taranto, e segnatamente della zona Tamburi, quel quartiere residenziale attaccato alla fabbrica e irresponsabilmente autorizzato negli anni all'espansione? Un inquinamento con conclamati danni alla salute dei lavoratori e dei cittadini, dovuto alle vaste aree scoperte di stoccaggio dei parchi minerali; un inquinamento dovuto agli altiforni e allo *slopping*, quel frequente fenomeno di dense ed enormi nubi rossastre uscenti dalle due acciaierie ormai diventato l'emblema negativo dell'impianto di Taranto. È mai possibile che solo i cittadini se ne accorgessero? L'Ilva è un gigante mostruoso, anzi un ecomostro, diventato tale per responsabilità della proprietà: prima lo Stato, sino al 1995, poi del privato. Ma l'Ilva è anche sinonimo di negligenza, di disprezzo ambientale e di noncuranza della salute pubblica anche per responsabilità e complicità degli enti come Comune, Provincia e Regione e degli organismi di controllo che non hanno vigilato: l'ASL, prima, e, dal 2003, l'ARPA Puglia. Questo succedeva mentre al Nord le nostre imprese vengono tartassate continuamente dagli enti di controllo. Per troppi anni è stato ignorato l'inquinamento diffuso della qualità dell'aria, del suolo e delle falde idriche, per troppi anni sono state omesse indagini epidemiologiche per verificare l'incidenza degli inquinanti. È dovuta intervenire la magistratura affinché le autorità preposte ai controlli si accorgessero che a Taranto si stavano compiendo illeciti ambientali con impatto gravissimo sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. È evidente che la proprietà dell'Ilva, negli anni, non ha destinato parte dei profitti per adeguare gli impianti alle prescrizioni dell'AIA, non solo alle migliori tecnologie disponibili, ma anche alle più elementari opere, ad eccezione delle rare installazioni fatte negli ultimi mesi, che per la verità sono pochissime e dunque riteniamo che non basteranno trentasei mesi di commissariamento. Sono infatti pressoché assenti le coperture dei nastri trasportatori e delle aree di stoccaggio dei minerali, mancano addirittura i sistemi di captazione polveri con i filtri. La risposta governativa all'iniziativa della magistratura è stata l'emanazione, negli ultimi undici mesi, di una raffica di frettolosi e approssimativi decreti‑legge

Il decreto-legge blindato che ci apprestiamo a convertire, oltre a non essere risolutivo, è pieno di elementi critici, per stessa ammissione del Governo e della maggioranza. con un ordine del giorno *omnibus* presentato nelle Commissioni riunite del Senato la maggioranza ha di fatto conferito una delega all'Esecutivo per affrontare i diversi nodi rimasti scoperti, fra i quali anche il finanziamento all'ISPRA e all'ARPA Puglia. alle Agenzie regionali del Nord? Niente? La Lega Nord condivide la scelta della prosecuzione dell'attività industriale, sia per salvaguardare i livelli occupazionali, sia perché solo così si autofinanziano gli interventi di risanamento ambientale. Condividiamo il principio secondo cui «chi inquina paga», e sono già state troppe le risorse pubbliche distolte. Non possiamo permetterci il fermo o la chiusura dello stabilimento, perché non vogliamo un'altra Bagnoli, un'area abbandonata e degradata, ma soprattutto non vogliamo rischi per la stabilità degli altri stabilimenti Ilva per la lavorazione a freddo situati al Nord, ovvero quelli di Genova, Novi Ligure e Racconigi. La Lega Nord, però, non approva questo decreto-legge, sia per diversi contenuti non condivisibili, sia per le sue profonde lacune. al commissariamento di tutta l'impresa Ilva, che è una novità rispetto ai due decreti precedenti. Con un nostro emendamento respinto dal Governo, che interpretava anche le richieste del mondo imprenditoriale, chiedevamo di limitare il commissariamento al solo impianto di Taranto, perché è solo qui che l'AIA, che è specifica per ogni stabilimento, è stata disattesa. del commissariamento anche agli altri stabilimenti Ilva, che non evidenziano inadempienze ambientali, rappresenta una lesione del diritto di proprietà, una prevaricazione nei confronti dei piccoli azionisti e un'interferenza con la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione.

di interesse strategico nazionale. È migliorativa, ma non basta, la modifica introdotta alla Camera dei deputati che, accogliendo gli emendamenti presentati da diversi Gruppi, compreso quello della Lega Nord, ha almeno previsto la possibilità di limitare il commissariamento al singolo stabilimento di imprese con almeno 1.000 lavoratori subordinati. Ribadiamo però che il decreto va comunque, anche in questo caso, a costituire un precedente pericoloso per l'attività economica privata. La peculiarità di Taranto, non assimilabile ed equiparabile ad altre situazioni esistenti nel Paese, avrebbe dovuto suggerire una scelta diversa, con un provvedimento specifico. Invece si è preferito conferire un potere discrezionale al Governo, nella scelta delle imprese da commissariare, introducendo di fatto, come qualcuno ha affermato, una nuova via italiana al socialismo. *(Applausi dal perché, nonostante l'occasione del decreto, non si vuole ancora una volta risolvere il problema dirimente dello smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività industriale e dalla bonifica. Un problema, quello della ruera (così la chiamiamo al Nord) che ritroviamo troppo spesso quando discutiamo di un territorio del Sud Italia. Eppure le discariche nell'area della fabbrica di Taranto esistono, con capacità di stoccaggio pari a diversi anni, già promosse nella valutazione di impatto ambientale, come ha anche affermato il subcommissario Ronchi, ma che per motivi a noi incomprensibili non sono state ancora autorizzate all'utilizzo. Abbiamo sollevato il problema con un nostro emendamento, ma Governo e maggioranza non hanno voluto accoglierlo, siamo certi per compiacere tanti, e in particolare la Regione Puglia e il suo Presidente.

oppure gravare di oltre 300 milioni il quadro economico dell'operazione, pensando di smaltire altrove i rifiuti. Ma qui scordatevi di dirottarli al Nord. *(Applausi al decreto perché respingendo un nostro emendamento si ufficializza un palese conflitto di interesse, consentendo che a fare il commissario straordinario possa essere chiamato un precedente amministratore, che non può non avere corresponsabilità nelle inadempienze relative all'AIA. Diciamo infine no perché il decreto‑legge prevede una speciale deroga al Patto di stabilità per la Regione Puglia. una palese disuguaglianza fra i territori: non possono esserci figli e figliastri, visto che emergenze analoghe ed esigenze di vario tipo ci sono anche nelle Regioni per le quali la facoltà di deroga viene sempre preclusa. PRESIDENTE. La invito

Come detto, quello in votazione non sarà l'ultimo provvedimento per Taranto. Tra pochissimi mesi si dovrà trattarne un quarto, un decreto ministeriale, per dare risposta ai problemi che oggi irresponsabilmente lasciamo senza soluzione. Ci domandiamo se un *poker* di decreti basterà. Noi della Lega Nord ne dubitiamo fortemente, così come dubitiamo che Taranto potrà rappresentare un modello di riferimento per il settore siderurgico anche in Europa. L'approccio al problema è partito con il piede sbagliato e prosegue in peggio. Per tutte le ragioni sopra esposte, a nome del Gruppo Lega Nord e Autonomie, comunico il voto fortemente negativo sul provvedimento.

onorevoli colleghi, non leggerò il testo dell'intervento che avevo preparato, perché penso che Taranto abbia bisogno di più rispetto e generosità da parte di quest'Aula. di quest'Aula. Al danno che oggi ha Taranto abbiamo contribuito tutti: quelli che erano in questo Parlamento, quelli che erano fuori, i cittadini di quel territorio che hanno visto fare e non hanno detto nulla, quelli che fino a qualche tempo fa erano nelle amministrazioni comunali, provinciali e regionali di quel territorio. In questo Parlamento continuo a vedere il Nord contro il Sud, la destra contro la sinistra,

chi ci ha mandato qui, chi ci ha dato questa delega. Ho avuto una vita che mi ha premiato molto, mi ha portato in giro per il mondo, mi ha fatto sedere in tanti posti importanti, eppure da quando sono qua sono sempre molto emozionata, perché in giro per il mondo rappresentavo me stessa, il mio gruppo, le persone che erano con me, invece qua rappresento i cittadini di questa terra.

È inutile venire qua e dire che siamo tutti belli e puri. Noi oggi stiamo affrontando una nuova sfida; stiamo commissariando un'azienda privata. Stiamo spiegando agli imprenditori italiani che è finito il tempo in cui facevano quello che volevano ed è arrivato il tempo di seguire le leggi, perché queste esistono già. Noi forse non dovremmo nemmeno convertire altri decreti per fare queste cose, ma dobbiamo fare in modo che tutti gli operatori che tutti gli operatori di questo Paese seguano le leggi. In quest'Aula, tra ieri e oggi, ho sentito tante cose, anche tante belle favole, senza la fine però. però. Nelle favole bisogna mettere la fine. C'è chi vuole chiudere l'impresa perché fa 1.600 morti, però forse nessuno si rende conto di avere ai piedi un paio di scarpe

quindi, che il rispetto e l'etica ci fosse in tutto il mondo. Se noi siamo veramente quello che vogliamo raccontare alle persone, se vogliamo essere quello che continuiamo a dire in quest'Aula, secondo me, dobbiamo

senatrici e senatori, so che molti di voi voteranno per appartenenza politica, anche i colleghi pugliesi del "partito unico", nonostante le decine di audizioni chiarissime nei contenuti

di descrivere perché il Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle voterà contro questo disegno di legge descrivendolo non a voi, che avevate già deciso come procedere prima e a prescindere da ogni approfondimento fatto, ma a chi segue i lavori del Senato da casa e ha speranza di verità e giustizia. In questa dichiarazione di voto contrario userò molte parole non mie, perché tante verità sono già state scritte nei mesi scorsi e meritano di essere riportate in quest'Aula. Dichiaro il voto contrario perché è confermata l'abrogazione della figura del Garante per l'attuazione delle prescrizioni, introdotta con la legge n. 231 del 2012 dal Governo Monti. Ora sarà lo stesso commissario Bondi, d'intesa con Regione ed enti locali, a fornire ai cittadini «dettagliatissime» e «continue» informazioni sul reale andamento delle operazioni di risanamento all'interno dell'Ilva. Figuriamoci! Dichiaro il voto contrario perché il rapporto di valutazione del danno sanitario, introdotto da una specifica legge della Regione Puglia la scorsa estate, non potrà modificare le prescrizioni dell'AIA: ovvero viene cancellato l'unico motivo per cui quella legge avesse un senso. la decisione non poteva essere diversa, dopo che il 29 maggio scorso Giorgio Assennato, direttore di ARPA Puglia, ha illustrato il rapporto elaborato nell'ambito della valutazione del danno sanitario. In 99 pagine di studio, Assennato sostiene infatti - e qui cito - che «i miglioramenti delle prestazioni ambientali, che erano conseguibili con la completa attuazione della nuova AIA (...), comportano un dimezzamento del rischio cancerogeno della popolazione residente intorno all'area industriale». Dichiaro inoltre il voto contrario perché, nonostante sia previsto l'allentamento del Patto di stabilimento interno della Regione Puglia per favorire le azioni di bonifica, per cui l'ente potrà sforare il Patto per 1,3 milioni nel 2013 e per 40 milioni nel 2014 (per le spese necessarie agli interventi previsti), i calcoli non tornano per nulla, perché il protocollo firmato il 26 luglio dell'anno scorso prevedeva fondi stanziati per 119 milioni. Lo sforamento di fondi per 41,3 milioni sino al 2014 non potrà mai garantire l'adeguata copertura per gli interventi previsti, che ammontano nel dettaglio a: 40 milioni 21 milioni per la bonifica e messa in sicurezza permanente dei sedimenti contaminati da PCB nel Mar Piccolo; altri 50 milioni di euro per la messa in sicurezza e bonifica della falda superficiale; infine, 8 milioni per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere

ha scoperto le carte di quello che è il senso vero del gigantesco inganno celato da questo disegno di legge, affermando - e qui cito ancora - che «si sta predisponendo un piano finanziario che, attraverso una negoziazione con le banche e la BEI, metterà a disposizione 1,8 miliardi di euro in tre anni per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'AIA». Dunque, come preannunciato da alcuni negli ultimi mesi, non solo il gruppo Riva non scucirà un euro per il risanamento degli impianti e dell'area a caldo, ma non lo farà neppure Ilva SpA. Del resto, erano già in tanti a denunciare come Ilva SpA non disponga delle risorse finanziarie per espletare anche una sola delle prescrizioni più importanti inserite nell'AIA, tanto che il responsabile delle relazioni esterne di Ilva, dottor Martino, ebbe a spiegare qualche giorno fa ai sindacati - e qui cito di nuovo - che «le risorse generate dall'attività industriale bastano soltanto per pagare stipendi, materie prime e fornitori». Stando così le cose, è molto probabile che siano state le stesse banche e la Banca europea per gli investimenti ad indicare il signor Enrico Bondi come l'unica persona adatta a ricoprire l'incarico di commissario, con il Governo che si è dovuto piegare, pur sapendo di palesare alla luce del sole un conflitto di interessi macroscopico, visto che lo stesso Bondi era stato nominato dalla famiglia Riva, soltanto ad aprile scorso, come amministratore delegato dell'Ilva SpA. Presidente, io credo che non ci voglia molto per districarsi tra le contraddizioni odierne della città di Taranto, che si incarnano nel conflitto tra due diritti inalienabili, quello al lavoro e quello alla salute, quest'ultimo condizionato dall'ambiente.

dai quali io traggo la considerazione che le responsabilità della distruzione ambientale e del conseguente disastro che colpisce operai e cittadini di Taranto non potranno mai essere equamente divise tra chi impone un ricatto e chi talvolta è costretto a subirlo perché è debole e viene afferrato alla gola da chi usa tutto il suo potere per cancellare il riscatto insito nella cultura del lavoro. Se è vero che chi fa impresa ha il diritto di garantirsi degli utili, è altrettanto vero che i profitti non possono e non devono essere accumulati a danno di chi lavora e della collettività. Ma questo non è ciò che appare o che si vuole far apparire, visto che si ripropone ancora una volta la teoria dei due interessi contrapposti: da un lato, quello delle maestranze dell'Ilva che difendono il loro lavoro ad ogni costo, anche se il prezzo da pagare è un tumore al polmone e l'inquinamento del territorio; dall'altro, quello dei cittadini che mettono al primo posto la salute, in nome della quale pretendono la chiusura del più grande stabilimento siderurgico d'Europa, o almeno della sua area a caldo. Ma che idea della cittadinanza è questa che esclude gli operai? Persino una parte dell'ambientalismo più sensibile alla condizione operaia pretende da loro l'obiezione di coscienza, cioè il rifiuto di lavorare se il prodotto della propria attività provoca un danno sanitario a sé e alla collettività. Così, nella latitanza o, peggio, con la complicità di tanta politica e tante istituzioni pubbliche e private, laiche e religiose, di tanta stampa e di parte dei sindacati asserviti al padrone, si perde di vista il nemico principale, il padrone appunto, che grazie a tanta subalternità è riuscito a scatenare la guerra tra poveri, tra le vittime della sua avidità, trasformando il conflitto classico tra capitale e lavoro in un conflitto tra pari: pari, però, nella disgrazia e nel dolore. Poiché però l'ingiustizia sociale riflette l'ingiustizia ambientale, quando una fabbrica inquina, i suoi veleni ammazzano anzitutto chi lavora dentro quella fabbrica; poi devastano il territorio dove è collocata, che raramente è un quartiere delle *élite* urbane, e fanno ammalare chi ci vive; ed infine i suoi scarti trovano la via che li condurrà in qualche discarica del sud del mondo o magari di quei tanti sud dove vivono i poveri del nord. Il conflitto tra i diritti fondamentali al lavoro e alla salute ha una storia lunga, che inizia ben prima dell'Ilva di Taranto. Viene da lontano, dagli impianti chimici di Porto Marghera, dall'ACNA di Cengio, da altri impianti inquinanti in Liguria, in Puglia, in Toscana, in Campania. Viene da Casale Monferrato, dove decenni dopo la chiusura della Eternit si continua a morire di mesotelioma. Ma all'Ilva questo conflitto ha una specificità che si chiama Emilio Riva, il "rottamaio": colui che con quattro soldi si è portato a casa la siderurgia italiana svenduta dallo Stato che, invece di tutelare un bene della collettività, ha scelto di liberarsene, incassando per questa tipica privatizzazione all'italiana la metà dei soldi spesi per ammodernare lo stabilimento tarantino. Quando però finalmente a Taranto si materializza la percezione del disastro ambientale e sanitario provocato da diossina, PCB, polveri sottili e metalli pesanti, comincia a svilupparsi una sensibilità prima ambientalista e poi anche economica. Riva, grazie ad un utilizzo senza precedenti della legge sull'amianto, svuota la fabbrica mandando a casa 12.000 lavoratori cinquantenni chiamandoli usurati, per sostituirli con altrettanti giovani meno costosi. Oggi, finalmente, tante persone si sono convinte di una cosa: Riva è ormai incompatibile con Taranto, e forse persino con l'intera siderurgia italiana. Io ho provato a capire se una diversa Ilva sia ancora compatibile, e a quali condizioni, con Taranto. Probabilmente l'unica strada per tentare di salvare lavoro, economia e salute sarebbe quella di liberarsi di chi si è reso responsabile del disastro di Taranto, facendogli pagare interamente e da tutti i punti di vista i costi

per la prima volta nel nostro Paese e, quindi, nel nostro ordinamento, l'istituto del commissariamento straordinario di un'azienda privata per l'ottemperamento a prescrizioni normative in materia ambientale trova allocazione. Conosciamo le vicende economiche, sociali e giudiziarie che da qualche anno interessano lo stabilimento dell'Ilva di Taranto. È una collettività fortemente preoccupata del territorio di Taranto che, se da un lato ha beneficiato delle ricadute occupazionali derivanti dalla presenza di un complesso industriale e siderurgico tra i più significativi d'Europa, dall'altro ne ha sopportato le conseguenze negative in termini di impatto ambientale e sanitario. Ma qui c'è anche un'altra questione, Presidente. Dobbiamo porci l'interrogativo di quale possa essere il presente ma soprattutto il futuro del nostro Paese, un grande Paese. La prima domanda da porci è se può esistere un grande Paese senza un grande apparato industriale. Questo è un argomento fondato. E un grande apparato industriale

punto una tematica, quella dell'interesse nazionale che, evidentemente, in un caso di questo genere si deve bilanciare con altri diritti costituzionalmente garantiti: il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto d'impresa, la libertà d'iniziativa economica e anche il dovere da parte di tutti noi di salvaguardare l'ambiente. Peraltro, risulta evidente la forte incisività con la quale si va a gravare sull'autonomia privata e sui contenuti della libertà economica, intesa come principio politico e come diritto individuale, libertà che subisce una significativa compressione con la disciplina generale ed astratta del commissariamento disposta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013. È pertanto all'esame dell'Assemblea del Senato un'applicazione paradigmatica del principio sancito dall'articolo 41 della Costituzione che recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Va quindi osservato che la limitazione della libertà di iniziativa economica è, in queste circostanze, giustificata dall'impellente necessità di approntare rimedi urgenti alla compromessa situazione ambientale. Nel riflettere sui rapporti intercorrenti tra il principio di libertà del comma 1 dell'articolo 41 della Costituzione ed il limite dell'utilità sociale contenuto nel comma 2 dello stesso articolo, ritengo che i limiti imposti dall'esigenza di garantire la sicurezza, la libertà e la dignità umana rappresentino, pur sempre, limiti esterni esterni all'attività economica privata. Tali limiti vengono assunti nel contesto di una maturata consapevolezza delle conseguenze sanitarie e di una responsabilità ambientale rispetto alla collettività interessata ed alle generazioni future della città di Taranto e dei territori limitrofi. Il sopralluogo allo stabilimento dell'Ilva di Taranto effettuato da una delegazione delle Commissioni riunite ha consentito di acquisire maggiore consapevolezza delle particolari complessità di un contesto ambientale, economico e sociale e una più forte determinazione del Parlamento nell'intenzione di risolverle. Il decreto-legge che oggi convertiamo è quindi importante perché affronta, a nostro avviso in materia equilibrata, una situazione di conflitto che si è venuta a creare tra problemi ambientali, problemi di salute e problemi di lavoro. Pure nel contesto della crisi in cui si trova oggi l'economia italiana, l'Ilva di Taranto significa una capacità occupazionale di circa 12.000 unità che, con l'indotto, divengono 20.000,

Il decreto individua nel commissariamento lo strumento più idoneo per arrivare a superare le inottemperanze all'AIA in tempi certi e garantisce che il prosieguo dell'attività di impresa possa mantenere il livello occupazionale, generando quelle risorse necessarie perché le inottemperanze all'AIA possano essere superate e possa essere assicurata la qualità ambientale, la riqualificazione e soprattutto l'occupazione dei cittadini. Ciò rappresenta una garanzia per il sistema Paese, perché non deve essere posta in discussione la capacità d'impresa, il diritto d'impresa e dell'attività privata. Per quanto concerne gli aspetti che riguardano gli interventi finalizzati alla prevenzione ambientale e sanitaria, si sottolinea l'introduzione di esperti in materia di salute, ambiente e attività industriale, che hanno il compito importante di verificare e garantire il piano di azioni necessarie per il rispetto dell'AIA.

si ricorda ancora che, per la prima volta, si prevede il commissariamento per motivazioni ambientali e si prevede altresì l'assunzione, da parte della struttura preposta al commissariamento, della responsabilità dell'intero governo del processo produttivo. Il decreto-legge è inoltre basato sull'assunto che i cittadini e, con essi, il bilancio dello Stato non devono farsi carico di responsabilità economiche che rimangono e devono rimanere in capo all'impresa. Al commissario compete l'onere di adottare tutte le azioni utili a tutelare l'ambiente e la qualità della vita nei contesti nei quali si sviluppa l'attività produttiva di imprese definite strategiche e che, strategiche, lo sono veramente, nella piena consapevolezza che una interruzione della produzione potrebbe arrecare gravi danni all'economia nazionale, oltre che all'ambiente e alla salute degli abitanti e delle comunità interessate. Signor Presidente, ci troviamo di fronte l'esempio di un decreto che nasce da motivazioni fondate e che rappresenta una sperimentazione importante nel nostro Paese ed abbiamo la consapevolezza, questa volta, che il legislatore e il Parlamento hanno ben operato, tenendo ben presente l'equilibrio tra i vari diritti costituzionali che devono essere garantiti. Ed è proprio per queste ragioni che il Popolo della Libertà preannuncia convintamente il proprio voto favorevole.

il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare è innanzitutto un atto dovuto e non più procrastinabile che testimonia, dopo il buon intervento della magistratura, il coraggio di questo Governo nell'affrontare una problematica - e mi riferisco in particolare alla grave situazione dell'Ilva di Taranto - caratterizzata da decenni di errori, assenze e dimenticanze e sfociata nella drammatica contrapposizione tra necessità d'impresa e tutela dei diritti. La vicenda dell'Ilva, così come quelle legate a molte altre realtà industriali italiane, palesa in maniera drammatica la contraddizione e il fallimento, ancor più evidenti in un contesto di grave crisi economica, di un sistema produttivo che per decenni ha anteposto l'esigenza di garantire la produzione, e con essa anche il lavoro e il massimo profitto, alla necessità di tutelare la salute del cittadino e di salvaguardare l'ambiente, diritti fondamentali di ogni cittadino, nei confronti dei tali né gli amministratori delle aziende interessate, né la classe politica hanno saputo fornire per tempo risposte adeguate, quasi fosse impossibile garantirli senza determinare effetti devastanti sull'attività produttiva e quindi sull'occupazione. Credo innanzitutto che sia doveroso ricordare di cosa stiamo parlando: ovvero di cinquant'anni di storia industriale del nostro Paese. Quando, nel 1961, Taranto fu scelta per ospitare il quarto e più grande polo siderurgico italiano, la società pubblica Italsider rappresentava rappresentava un'eccellenza non solo nel panorama italiano, ma anche in quello europeo. Lo stabilimento, per circa un ventennio, è stato protagonista di un forte sviluppo produttivo, all'avanguardia e capace di primeggiare con prodotti innovativi con i *competitor* internazionali, diventando il principale fornitore di materie prime delle migliori industrie metalmeccaniche mondiali e trascinando il miracolo economico italiano di quegli anni. Ancora oggi, nonostante la grave crisi economica che sta attraversando il settore siderurgico - come hanno ricordato ieri i relatori Tomaselli e Bruni, a cui va il mio ringraziamento - l'Ilva rappresenta una capacità occupazionale di circa 11.000 unità che, se sommate all'indotto, raggiungono le 16.000, il 75 per cento del PIL della provincia di Taranto e il 10 per cento del PIL della Puglia (come ricordato dal senatore Marinello). Stiamo parlando della più grande acciaieria d'Europa, con una capacità produttiva di 9-10 milioni di tonnellate annue prodotte, pari al 57 per cento della produzione totale in Italia, e con un'estensione di 1,5 milioni di metri quadrati e un parco minerario all'aperto di 78 ettari. Numeri che fanno girare la testa, cari colleghi. Ora, ben consapevoli di quanto la dismissione di un sito inquinato possa essere anche peggiore della prosecuzione della sua produzione, il cui costo di bonifica e risanamento sarebbe interamente a carico dello Stato, non possiamo essere così miopi da decidere di privare il nostro Paese e Taranto di una realtà così importante. È una questione strategica: chiudere l'Ilva significa abbandonare l'industria siderurgica nazionale, con le conseguenti gravi ripercussioni sugli altri settori produttivi, primo fra tutti quello della meccanica. Anche dall'Europa emerge oggi l'indicazione chiarissima di tornare a produrre e ad investire nell'industria. Consci del ruolo cruciale che riveste il comparto siderurgico per l'industria europea, in un momento di crisi e di difficoltà, lo scorso 11 giugno europea ha infatti approvato un Piano di azione per l'acciaio, che indica la sostenibilità ambientale e l'innovazione tra le sei aree d'intervento su cui investire. Sostenibilità ambientale e innovazione: sono questi i presupposti da cui partire per un programma di sviluppo e di risanamento rigoroso, capace di produrre ricadute positive sull'ambiente, la salute e l'occupazione, non solo per l'Ilva, ma per tutte le numerose realtà produttive italiane. Taranto, infatti, non è solo Ilva, ma anche cementifici, raffineria, arsenale, centrali elettriche: un intero comparto industriale che, grazie al provvedimento in esame, potrebbe rilanciarsi e tornare a nuova vita. È quasi automatico per me fare una parallelismo con La Spezia, la mia terra, che ha davvero molto in comune con la cittadina pugliese, ma è un paradigma che può e deve essere esteso a tante altre realtà presenti sul nostro territorio, perché produrre salvaguardando la salute

per l'intero complesso produttivo italiano. Le modalità con cui saranno attuate le prescrizioni dell'AIA potranno generare un *know-how* da esportare, soprattutto se consideriamo che a distanza di 40 quarant'anni questo stabilimento ha bisogno di un costante ammodernamento. Innovazione, sostenibilità e cooperazione tra i vari siti produttivi dovranno essere le direttive da seguire, specializzandosi sempre più in quei comparti dove rappresentiamo l'eccellenza, come le opere infrastrutturali, la cantieristica navale, le *automotive* e le grosse tubazioni. L'attuazione dell'AIA, così come è stata declinata nelle sue prescrizioni, è in grado, se effettuata completamente e nel rispetto della tempistica indicata, di assicurare compiutamente la tutela dell'ambiente, ovvero di rendere sostenibile il processo produttivo dell'Ilva. Per questo motivo segnalo la necessità di garantire che, in sede di redazione del Piano strategico, non siano adottate modifiche all'AIA meno rigorose e stringenti rispetto a quelle vigenti o alle procedure previste dalla normativa nazionale.

ho avuto modo di esprimere personalmente al dottor Enrico Bondi il mio pensiero, che vorrei ribadire in questa autorevole Aula. Confermando l'apprezzamento per la figura e le competenze del commissario, mi preme sottolineare quanto l'incarico che si appresta ad eseguire sia delicato e importante. Tra i suoi compiti, infatti, non c'è solo quello di risanare un'azienda d'interesse nazionale ma, soprattutto, la grande responsabilità di contribuire a ricucire la profonda lacerazione del tessuto sociale che questa vicenda ha prodotto nella città. Quest'ultimo tema non può essere sottovalutato. Il commissario dovrà ascoltare e condividere, laddove è possibile, le voci del territorio, *in primis* Regione e Comune. Sono sicuro che da questo non potranno che scaturire utili benefici anche per il futuro dell'azienda. D'altra parte, la migliore risposta a Taranto, come altrove, saranno i fatti. Per quanto riguarda, invece, l'eliminazione della figura del Garante, che qui ha suscitato scandalo, possiamo comunque ritenerci soddisfatti della scelta di Edo Ronchi come subcommissario che affiancherà, nello svolgimento della sua funzione, il commissario Bondi con un ruolo esplicitamente rivolto all'ambientalizzazione a cui l'azienda deve prestare la massima attenzione. Edo Ronchi, per la sua storia e per le sue alte competenze, rappresenta una garanzia per dare credibilità al percorso di risanamento previsto dal decreto-legge e per contribuire a costruire un rapporto più forte con la città con la città e le sue istanze. Per i motivi appena elencati confido che gli stessi, commissario e subcommissario, in coerenza con le prescrizioni dell'AIA, saranno perfettamente in grado, sentite la Regione e l'ARPA, di individuare le migliori modalità per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo da proporre al Ministero dell'ambiente per l'emanazione dell'apposito decreto. Il decreto-legge, colleghi senatori, ha certamente ancora margini di miglioramento. Non mancano, infatti, punti su cui avremmo voluto dare un contributo, come ha ricordato nel suo ottimo intervento il senatore Mucchetti, ma l'allungamento dei tempi dell'esame di altri provvedimenti, sia alla Camera dei deputati che al Senato, ha causato un pesante ingolfamento dei lavori parlamentari e l'impossibilità di una terza lettura del disegno di legge in tempo per la convenzione del decreto-legge, che scade Tutto questo, colleghi senatori, ci investe di una grande responsabilità: quella di non far decadere un provvedimento così importante che segna un punto di svolta nel rapporto tra esigenza produttiva, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e tutela della salute, tematiche ormai non più prorogabili. Il Partito Democratico nell'aver assunto anche questa responsabilità non ha nulla di cui vergognarsi, colleghi senatori. È questa oggi la sfida per chi vuole governare il territorio, senza demagogia e proclami inattuabili e senza raccontare favole, ma con il coraggio necessario a far sì che, tenendo conto degli errori del passato, con responsabilità si possano attuare politiche giuste, innovative e rispettose dei diritti fondamentali dell'uomo, consentendo a questa parte dell'Italia di riappropriarsi del proprio futuro. L'Italia ce la può fare se riesce a riconoscere e a valorizzare i suoi fondamentali e le sue competenze, e vi assicuro che ne abbiamo molte. Per questi motivi dichiarato, a nome Gruppo parlamentare del Partito Democratico, il voto favorevole per l'approvazione, senza modifiche, del testo licenziato dalla Camera.

a intervenute esigenze del mio Gruppo di riunirsi urgentemente per analizzare le dinamiche e gli effetti di eventi che si sono realizzati stamani in occasione dell'elezione dei vertici di alcune Commissioni,

Signor Presidente, intervengo in merito alla soppressione della sezione distaccata del tribunale di Viareggio, per il quale è previsto l'accorpamento al tribunale di Lucca a partire dal settembre prossimo. Sono consapevole che la *ratio* del decreto legislativo n. 155 del 2012, che prevede la soppressione e il conseguente accorpamento di 31 tribunali e di 220 sezioni distaccate di tribunale su tutto il territorio nazionale, rientra nell'esigenza di razionalizzazione delle stesse e di riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, ma nel caso della sezione distaccata di Viareggio tale esigenza non si ravvisa, in quanto l'accorpamento al tribunale di Lucca comporterà una spesa per il Comune di Lucca di ben 3 milioni di euro. Considerato che il carico di lavoro maggiormente elevato nel penale, per quanto riguarda il tribunale di Lucca, ravvisa 1.683 procedimenti su 2.387, pari ai due terzi delle cause penali, e di pari entità nel civile, non si capisce proprio la *ratio* di questo accorpamento. Quindi, spero e mi voglio augurare che nel decreto del fare quantomeno venga approvato o considerato l'emendamento che prevede la proroga almeno di un anno della chiusura della revisione delle circoscrizioni giudiziarie

Signor Presidente, voglio portare alla vostra attenzione un caso di licenziamento ingiusto, che però è sintomatico di uno stato della Nazione. Come in tantissimi altri casi, è esemplare questo caso di licenziamento in un contesto terribile in cui si trovano oggi tantissimi lavoratori, soprattutto i lavoratori sindacalisti. Giuseppe Larobina, detto Pino, è stato licenziato dalla Kuehne Nagel (ex IVECO) di Torino con una scusa, senza che avesse mai subito un procedimento disciplinare. È stato licenziato solo per la sua attività sindacale di base. Per chi non lo sapesse in quest'Aula, gli USB sono sindacati fatti da lavoratori veri, non la casta CGIL, CISL e UIL. Sono lavoratori che usano il loro tempo libero per difendere i loro diritti e quelli dei loro colleghi e dei loro compagni di lavoro. Pino è stato mobbizzato, controllato, seguito addirittura da investigatori privati pagati dall'azienda per scoprire alla fine che lui usava i permessi sindacali per fare il sindacalista (pensate un po'), e nonostante ciò è stato licenziato. Questo stato di ricatto permanente ai lavoratori è inaccettabile, è diventato intollerabile. Io denuncio in quest'Aula le mille storie quotidiane uguali a quella di Pino, la violenza psicologica e le discriminazioni che subiscono e la totale assenza di qualsiasi garanzia e protezione dei lavoratori. L'Italia è diventata una nazione di schiavi! I partiti e i Governi hanno permesso l'azzeramento dei risultati ottenuti da una lotta sindacale centenaria. E meno male che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, altrimenti cosa avreste fatto?

Signor Presidente, c'è uno sdegno che è trasversale, uno sdegno che avrà un importante appuntamento davanti alla prefettura di Bergamo stasera, alle ore 18,30. I sindaci si troveranno per manifestare contro la sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittime le multe ai Comuni delle Regioni a Statuto speciale, in particolare quelli siciliani: Comuni che hanno sforato il Patto di stabilità, Comuni che hanno avuto una gestione inadeguata a quel principio del buon padre di famiglia da applicare quando si tratta di amministrare i Comuni. È assolutamente negativa la sentenza, signor Presidente: rende ancora più assurdo e insopportabile il disequilibrio tra i ruoli e i pesi che i Comuni virtuosi devono affrontare. I Comuni bergamaschi e più in generale quelli del Nord hanno sempre denunciato il capestro amministrativo del Patto di stabilità, ne hanno chiesto a più riprese e a gran voce l'eliminazione o almeno la rivisitazione per i Comuni virtuosi. Appunto, quelli virtuosi, signor Presidente, che si sono sentiti estremamente umiliati da questa sentenza: quelli che stanno predisponendo

problemi a stanziare risorse per asfaltare le strade, per i servizi sociali, per la sicurezza, e non certo per avere auto blu. La Lega Nord ha organizzato questa manifestazione chiamando a raccolta tutti i sindaci, di qualsiasi colore, e invita le altre Province del Nord ad organizzare uguali manifestazioni in tutto il Paese. È un rospo, signor Presidente, che gli amministratori non possono e non vogliono mandare giù, anche se tutto va giù, signor Presidente. Presidente, colleghi, 3 miliardi di euro - e sono tanti - è il costo di un'opera mai compiuta e che mai si dovrebbe fare. Parlo del corridoio A12- Appia, ovvero 100 chilometri di asfalto nuovi di zecca che andrebbero a depauperare ancora di più il territorio del sud-est dei Castelli romani, del sud-est di Roma. Quest'opera costerà 30 milioni di euro a chilometro per erigere una nuova, ennesima, inutile, grande opera. Grandi opere che non sono per il bene dei cittadini, ma esclusivamente per il bene delle tasche dei soliti noti.

Lo scherzetto della A12-Appia ci è già costato 100 milioni di euro in tredici anni, la costruzione di due società, una di seguito all'altra, con lo stesso consiglio di amministrazione, cioè l'ARCEA, poi destituita (solo questo passaggio è costato 43 milioni di euro per gli azionisti privati), e le autostrade del Lazio create *ad hoc* per un vergognoso solito nulla di fatto. Ministro e Governo forzano la Regione Lazio nei nefasti giochi di Sottile e Zingaretti, che hanno già deliberato una nuova discarica che taglia proprio le zone interessate anche da questa grande opera. Zone bellissime che sono già oggetto di progetti per inceneritori, centrali a biogas, discariche esistenti e in progettazione, cementificazione selvaggia, come quella del Divino Amore. Dicevo, si forza la Regione a presentare istanza per ottenere lo sblocco dal CIPE di altri 700 milioni di euro necessari per far fronte alla parte pubblica del progetto, inserito nel solito *projet financing* all'italiana: cioè, poca utilità e tante mazzette. Va cambiato il paradigma e una strada come la Pontina, che fa quasi 30 morti all'anno, deve essere messa in sicurezza e non fatta diventare autostrada: una bretella che andrebbe a devastare l'agricoltura, la nostra agricoltura di cui andiamo tanto fieri, in paesi che si mantengono con il settore agricolo, come Cori, Lariano, Velletri, Valmontone e Labico. Sarebbe la solita pura follia! Spesso ci dite: è l'Europa che ce lo chiede. Ecco, in questo caso l'Europa chiede di cambiare il paradigma degli spostamenti, non favorendo il trasporto su strada, peraltro già in forte crisi, ma migliorando il sistema dei mezzi pubblici che oggi nel Lazio sono al livello di terzo mondo, per chi li prende tutti i giorni. *(M5S)*. Un modello sostenibile vuol dire trasporto su rotaia. Voi pensate solo alla TAV Torino-Lione, ma non pensate ai treni locali. Bretelle, chilometri di asfalto, discariche, milioni di metri cubi di cemento e di inceneritori: questo è il vero terrorismo!